Dichiaro aperta la votazione.

L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

individuare bene il nodo istituzionale di questa fase politica della vita del nostro Paese. Abbiamo sottolineato la necessità di definire

nel nostro calendario provvedimenti molto importanti da esaminare, a cominciare da quello che discuteremo tra pochi minuti; ritengo però che il tema del rapporto fra Governo e Parlamento sia

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che l'articolo 30, comma 1, sia soppresso e che venga approvato 1'emendamento 30.500 (testo 2), sul quale il parere è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione del comma 4*-ter*; che all'articolo 30, comma 3, dopo la parola "istituito" siano aggiunte le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"; - che all'articolo 44, comma 1, dopo la parola "istituito" siano aggiunte le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"; che all'articolo 46 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; - che l'articolo 55 sia sostituito dal seguente: Agli oneri recati dall'articolo 19, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010,

e in euro 77.031.400 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 52.000.000 per l'anno 2009, euro 92.000.000 per l'anno 2010 ed euro 11.160.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione,

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1; b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2; c) quanto a euro 28.897.325 per l'anno 2009, euro 32.712.780 per l'anno 2010, 30.319.980 per l'anno 2011 e euro 53.876.500 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,

per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 19 e 39, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11*-ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"; - che la tabella n. 1 sia sostituita dalla seguente:

499.000 | 2.417.000 | 2.388.000 | | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 22.000 | 521.000 | 514.000 | | Ministero per i beni e le attività culturali | 526.000 | 1.971.000 | 1.947.000 | TOTALE | 48.401.000 | 64.795.000 | 56.886.000 | Esprime parere di semplice contrarietà in ordine all'articolo 51. Il parere è altresì reso con il seguente presupposto: - che alle attività di cui all'articolo 30, commi 2, 3, 4 e 5, in relazione alla tenuta dell'Albo ivi indicato, possa farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Sugli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.0.300, 8.0.301, 24.0.100, 31.100, 33.102, 33.101

54.0.302 e 55.500, nonché parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.101, 4.100, 4.103, 4.104, 48.305, 48.0.300. Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle seguenti proposte sulle quali il parere non ostativo è reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alle condizioni che seguono: che alle proposte 12.0.100 e 12.0.300, le parole: "per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010" siano sostituite dalle altre: "a decorrere dal 2009" e che le parole: "24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008" siano sostituite dalle altre: "22 dicembre 2008, n. 203"; che all'emendamento 32.0.100 (testo 2) siano soppressi i commi 10 e 13; - che alle proposte 33.0.102 e 39.0.100 la parola: "2008" sia sostituita dall'altra: "2009" e che le parole: "24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008" siano sostituite dalle altre: "22 dicembre 2008, n. 203"; che all'emendamento 39.106 il numero 4) della lettera *l)* venga soppresso.

Il Senato della Repubblica, considerate le l'ONG di assistenza e aiuto sanitario, Medici Senza Frontiere (MSF), conosciuta in tutto il mondo per il suo impegno umanitario, il 31 ottobre 2008 ha terminato la propria attività sull'isola di Lampedusa, per scadenza del protocollo di intesa stipulato con il Ministero dell'interno; Ministero dell'interno; MSF ha garantito dal 2002 visite mediche d'emergenza gratuite per i migranti che arrivano sull'isola dopo aver attraversato un drammatico viaggio in mare.

al servizio sanitario regionale; nei primi dieci mesi del 2008 le persone sbarcate sulle coste dell'isola di Lampedusa sono state più di 25.000; negli ultimi anni tra i migranti sbarcati a Lampedusa vi è stato un incremento di patologie dovute alle condizioni dei viaggi in mare (traumi, ipotermia, ustioni, rispetto agli anni scorsi la popolazione migrante è cambiata, dal momento che sempre più persone provengono da zone di guerra o Paesi colpiti da carestie, come Somalia, Eritrea, Sudan ed Etiopia (30 per cento); un dato rilevante è costituito dall'incremento del numero delle donne (12 per cento) e dei minori (8 per cento), con un aumento delle donne in gravidanza (151 dall'inizio dell'anno), impegna il Governo ad assicurare l'assistenza sanitaria alle popolazioni migranti anche attraverso la stipula di intese con le componenti medico-sanitarie presenti sull'isola di Lampedusa, ivi compresi Medici Senza Frontiere.

Presidente, la riformulazione dell'ordine del giorno va nel senso di sottolineare che l'azione di Medici Senza Frontiere è importante, ma non è l'unica che viene svolta sul fronte sanitario a Lampedusa. sanitario a Lampedusa. Il senatore Stiffoni si riferisce ad una parte dell'ordine del giorno che non è stata modificata dal Governo, su cui sinceramente in questo momento non sono in grado di rispondere e mi riservo di fornire delucidazioni dopo aver acquisito informazioni. a riconoscere il ruolo di Medici Senza Frontiere e a ricordare che non è l'unica realtà che opera su questo fronte.

Onorevoli colleghi, prima di passare all'esame degli emendamenti, avverto che, da parte del senatore Bianco e di altri senatori, è stata presentata la richiesta di sottoporre a scrutinio segreto diversi emendamenti ed articoli del disegno di legge all'ordine del giorno. Tale richiesta è stata annunciata ed illustrata dal senatore Casson nella seduta antimeridiana del 19 novembre 2008, a conclusione della discussione generale. La Presidenza, dopo avere attentamente valutato le richieste di votazioni a scrutinio segreto alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 113, commi 4 e 6, del Regolamento, precisa che le relative votazioni sono state ritenute ammissibili per gli emendamenti o gli articoli che introducono nuove fattispecie di reato ovvero operano modifiche alla disciplina di reati già previsti dall'ordinamento o disciplinano circostanze aggravanti o attenuanti (articoli 13, 25 e 27 della Costituzione); prevedono disposizioni concernenti la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (articolo 24 della Costituzione); recano modifiche al sistema delle misure di sicurezza e prevenzione, purché si traducano in restrizioni della libertà personale (articoli 13 e 25, terzo comma, della Costituzione); attengono al principio che la «responsabilità penale è personale» (articolo 27, primo comma, della Costituzione); riguardano i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (articolo 29 della Costituzione); incidono sulla tutela dell'infanzia e della gioventù (articolo 31 della Costituzione). La richiesta di voto segreto non è stata invece ritenuta ammissibile, per estraneità ai criteri sopra richiamati, sugli articoli 4 (acquisizione della cittadinanza), 5 (requisito della regolarità del soggiorno per il matrimonio dello straniero), 41 (accordo di integrazione per il permesso di soggiorno), 46 (concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio) e relativi emendamenti; nonché sugli emendamenti 18.0.300 e 18.0.301, concernenti le caratteristiche tecniche delle «bombolette» per difesa personale, 39.102, 39.800/1 e 39.118, sul pagamento di contributi per il permesso di soggiorno, 39.104 e 39.305, in materia di accesso alle prestazioni sanitarie, 39.306, sulla segnalazione all'autorità giudiziaria degli stranieri non in regola che accedono a prestazioni sanitarie. L'elenco degli emendamenti e degli articoli ammessi al voto segreto, nonché di quelli non ammessi, con le relative motivazioni, sarà distribuito ai Gruppi. La Presidenza ricorderà di volta in volta gli emendamenti e gli articoli sui quali è consentito lo scrutinio segreto, fermo restando che in ciascun caso la richiesta dovrà risultare sostenuta dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento. Infine, sono improponibili per estraneità alla materia trattata dal disegno di legge, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 01.101 (abrogazione della legge n. 124 del 2008 sulla sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato),

(modifica all'articolo 2630 del codice civile, in materia di sanzioni per mancate comunicazioni al registro delle imprese). Passiamo all'esame degli

a nostro modo di vedere assume un grande rilievo. Si parla della materia della sospensione della pena, ossia del beneficio che il giudice può concedere in caso di condanna dell'imputato ad una pena contenuta

nel valutare la possibilità di concessione del beneficio debba considerare gli elementi indicati all'articolo 133 del codice penale, ossia la condotta del reo, la reiterazione di condotte disdicevoli, il comportamento processuale, cioè una serie di parametri. Noi riteniamo che l'istituto della sospensione della pena vada

il beneficio della sospensione sul presupposto che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati - così stabilisce il primo comma dell'articolo 164 - debba rientrare anche

le risultanze desumibili dal servizio informatico previsto dall'articolo 97 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. non è altro che la previsione dell'inserimento

Questo archivio informatico, previsto dall'articolo 97 delle norme di attuazione, consente cioè di sapere se una persona sottoposta ad un processo è colpita da un'altra misura cautelare per altro reato, e se quella misura cautelare sia stata eseguita o meno. Sicché il giudice, nel valutare il giudice, nel valutare la meritevolezza del beneficio della sospensione, dovrà tener conto anche di questi dati espressamente previsti

non riusciamo a capire perché, nel concedere un beneficio che ha come presupposto il fatto che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati, il giudice non possa valutare anche questo elemento, ossia l'esistenza di altre misure cautelari per altri reati commessi. In questo modo, riteniamo che l'istituto della sospensione, che contiene un beneficio elargito più che concesso, rientri nei confini normali, ossia che ne possono beneficiare soltanto condannati

fase, nel corso del processo, di fronte a dati oggettivi ed anche a seguito di un processo di maturazione che spesso avviene grazie anche al supporto delle associazioni antiracket,

di un elenco di emendamenti di cui è prima firmataria la collega Della Monica, seguita dalle senatrici Vittoria Franco, Anna Serafini e tante altre colleghe del nostro Gruppo, che affronta una delle questioni che riteniamo debba vedere il Parlamento, a partire da questa Camera, cominciare a dare una risposta chiara: mi riferisco alle questioni dei maltrattamenti, delle molestie e dello *stalking.* Chiunque di noi abbia seguito, anche durante queste vacanze, le cronache quotidiane ha visto quanti episodi ci sono di donne che finiscono in ospedale, quando non direttamente uccise, il colpevole nel 90 per cento dei casi è il convivente o il fidanzato. Siamo di fronte a questa tipologia allarmante e nuova, che ci richiede anche uno sforzo normativo per cogliere la specificità della situazione di separati, divorziati, allontanati anche con provvedimento giudiziario, che hanno

della polizia e della magistratura di prevenire da un lato e di colpire seriamente dove necessario, e nemmeno di mettere in atto tutte quelle

La legge sulla sicurezza ha in sé la revisione di parti della legge sull'immigrazione, la revisione di parti consistenti del codice penale. Si affronta, cioè, in un unico testo di legge un insieme di partite molto vaste, ciascuna delle quali avrebbe richiesto, a nostro avviso, una riflessione separata ed organica. come ci siamo già chiesti quando abbiamo svolto il dibattito sul decreto sulla sicurezza - mi rivolgo al Governo - perché dobbiamo anticipare tutto in un provvedimento e non occuparci

La ministra Carfagna ha presentato un suo testo, che non è tra le priorità di questo Governo. Diamo allora un segno alle donne italiane e cominciamo, a partire da questo emendamento, ad occuparci anche di tale questione perché la sicurezza delle donne italiane è un bene prezioso tanto quanto il patrimonio degli italiani.

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile». Si applica la disposizione dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288».

proposta di stralcio S1.100 è favorevole e ne illustro le ragioni. Le modifiche dell'articolo 648-*bis* del codice penale introdurrebbero per la prima volta nel nostro ordinamento positivo la figura del reato del cosiddetto autoriciclaggio.

Tali proposte, inserite dalle Commissioni nel testo oggetto dell'odierna discussione, dovrebbero essere più opportunamente trattate in una sede apposita, per ragioni che in sintesi espongo. Una norma incriminatrice del cosiddetto autoriciclaggio necessita di approfondimenti per armonizzarla con la disciplina dettata in sede comunitaria. disegno di legge n. 231 del 2007, impone infatti l'individuazione di strumenti volti a perseguire le attività illecite di investimento anche all'estero e nel rispetto dei principi basilari programmatici imposti dalla convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio. Inoltre, lo stralcio si rende opportuno per problemi di coordinamento di diritto interno, ovvero per rendere coerenti le possibilità di modifiche normative in materia con l'intero sistema sanzionatorio penale di settore, in particolare con la normativa sulla circolazione del denaro contante, sulla segnalazione delle operazioni sospette e sui pagamenti con moneta elettronica, che imporrebbero l'adozione, auspicata anche dal governatore della Banca d'Italia lo scorso anno, di un codice unico della normativa antiriciclaggio, attualmente frammentaria e disorganica.

il motivo specifico di questa soppressione concerne il fatto che con un tratto di penna lineare e non adeguatamente motivato, veniva proposta dal Governo una modifica molto profonda della normativa concernente il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, così come formulata all'interno del codice penale.

una proposta di legge, Atto Camera n. 952, che affronta esattamente tali tematiche. Credo che nel rispetto necessario tra i due rami del Parlamento non sia il caso di sovrapporsi ad una materia che già in questo momento è istruita ed approfondita presso la Camera di deputati.

a titolo di misura di sicurezza dal codice penale alle norme di attuazione del codice di rito processuale penale. I nostri subemendamenti mirano a correggere la rubrica dell'articolo 183-*ter* nella misura in cui non richiama quali destinatari dell'allontanamento in questione anche i familiari dei cittadini dell'Unione europea. Non mi sembra una norma particolarmente

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è di grande attualità, come abbiamo sentito anche in inizio di seduta, il dibattito tutto politico sul ruolo del Parlamento rispetto alle iniziative e alle proposte del Governo e viceversa. Vorrei rilevare che questo è un esempio, non dei principalissimi e tuttavia non irrilevante, della positività della collaborazione tra Parlamento e Governo nell'arrivare a un punto di incontro di tipo normativo che, a mio parere, sintetizza abbastanza felicemente le varie istanze che possono essere proposte.

Non ignoro infatti che diversi colleghi, anche autorevolissimi giuristi, non sono di principio favorevoli alla reintroduzione di questo reato di oltraggio, per argomenti in verità tutt'altro che ignobili, anzi significativi; tuttavia, ve ne sono di notevoli, anche nuovi, che militano invece a favore della reintroduzione di un simile reato. Debbo ricordare però che la collaborazione tra Governo e parlamentari (in particolare ne debbo dare atto al collega Saltamartini che si è fatto promotore di varie proposte al riguardo, poi vi sono stati alcuni miei modesti interventi in Commissione ha portato ad una formulazione decisamente accettabile, perché torna al reato di oltraggio ma lo focalizza, lo circoscrive e lo circostanzia dal punto di vista soggettivo ed oggettivo. In altre parole, essa prevede nell'economia del reato, perché esso si possa concretizzare, il requisito del luogo pubblico o aperto al pubblico, (circostanza oggettiva), la presenza di più persone (anch'essa circostanza oggettiva), l'offesa dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (circostanza (circostanza temporale oggettiva ed anche soggettiva), dunque della persona non solo in quanto tale, ma in quanto sta esercitando le sue funzioni, e che riceva l'offesa all'onore e al prestigio in quanto ed a causa delle sue funzioni.

forense - sull'onere della prova, sul fatto di non rimettere all'indiscriminata, ancorché pregevole asserzione del pubblico ufficiale che si asserisce offeso. La presenza di più persone, di per se stessa comporta la possibilità di una prova in termini di intervento testimoniale di soggetti che possano avere assistito al fatto oltraggioso. Mi sembra che la riformulazione, che nasce - lo ripeto - dalla collaborazione tra Governo e Parlamento nei suoi vari settori, sia un esempio classico di positiva collaborazione tra esecutivo e legislativo, che può portare a mio parere - tutte le norme sono criticabili, per carità - a un equilibrio delle esigenze rappresentate dalla norma e dei beni tutelabili decisamente apprezzabile. Con tutto il rispetto di principio per coloro che non condividono la sussistenza del reato come tale in via generale, milito a favore della positività di questa soluzione e mi esprimerò con voto favorevole alla formulazione sottopostaci dagli onorevoli relatori. Signora Presidente, intervengo per aderire alla richiesta formulata dal relatore per il ritiro dell'emendamento 1.200 ma soprattutto per sottolineare l'importanza e la svolta storica che oggi, con questa votazione, il Parlamento della Repubblica compie in merito alla tutela istituzionale delle forze di polizia. polizia. Avevamo inserito nel programma di Governo una più efficace tutela dell'azione delle forze dell'ordine e l'abbiamo realizzata con il decreto-legge n. 92 del 2008, reintroducendo il reato di ergastolo per l'omicidio di appartenenti alle forze dell'ordine. Con tale emendamento reintroduciamo il reato di oltraggio nei riguardi della funzione degli operatori delle forze dell'ordine e credo che in tal modo compiamo una svolta culturale sul piano giuridico e di politica del diritto una volta per tutte, comprendendo che la tutela della dignità delle funzioni delle forze dell'ordine e delle istituzioni nel nostro Paese meriti la protezione di norme penali incriminatrici. Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono davvero onorato, essendo stato per 32 anni un appartenente alle forze dell'ordine, di aver presentato questo emendamento, che spero entrerà a fare parte

di omicidio di appartenenti alle forze dell'ordine, nonché il reato di oltraggio nei riguardi delle forze di polizia. Dalla politica delle chiacchiere, dalla richiesta della Commissione d'indagine sui fatti di Genova contro le polizie ad una politica del diritto di tutela delle istituzioni dello Stato.

Ricordo semplicemente che il riferimento è alla norma di cui all'articolo 376 del codice penale, che riguarda la possibilità di considerare non punibile una persona che ritratta relativamente a tutta una serie di reati.

quindi che le indicazioni dei Presidenti delle Commissioni riunite, così come era maturata l'idea all'interno delle Commissioni stesse, possano essere un segnale positivo positivo di un Parlamento e di un Senato, in particolare, che congiuntamente vota una norma a sostegno della lotta contro la criminalità, con specifico riferimento al reato di estorsione.

subiscano una rivisitazione da parte degli autori possono essere dichiarati non punibili, estendere la gamma di queste possibilità, e limitarla nello stesso tempo, crea un disagio costituzionale di tutta evidenza. Capisco che per ogni reato, parlo in linea teorica, chiunque abbia rassegnato delle falsità agli inquirenti possa ritrattare ed essere dichiarato non punibile, ma per talune vicende particolari, se è certamente commendevole il principio - per l'amor del cielo, nessuno discute l'apprezzabilità delle ragioni - il dato costituzionale, Presidente, a mio avviso è ineludibile. Per questa ragione credo che l'Aula dovrebbe riconsiderare le argomentazioni dottamente introdotte dai colleghi che mi hanno preceduto sul tema e cercare di non vulnerare il sistema esprimendo

prevede la possibilità di estendere all'ipotesi del favoreggiamento quanto previsto per la falsa testimonianza. Pertanto, la sua preoccupazione, che in teoria

attinenti al provvedimento che stiamo discutendo; mi chiedo cosa ci sia di più attinente del contrasto alla violenza sulle donne che si esercita in luoghi pubblici, oltre che in famiglia.

proponiamo che venga introdotta la inescusabilità dell'ignoranza dell'età della persona offesa. È vero che alla Camera sono già all'ordine del giorno misure come quella inerente lo *stalking* e il provvedimento sulla violenza sessuale,

segnali chiari, evidenti e trasparenti di misure per il contrasto alla violenza sulle donne?

hanno una grande rilevanza e non credo che l'abbiano solo per le parlamentari donne. Penso che oramai sia evidente

segnala un'evidente crisi in termini di sicurezza nei rapporti interpersonali. C'è sempre un provvedimento più avanti, più urgente, più rapido, e questo è uno di quelli, ma ritengo che la sede più propria che possa ricomprendere in un testo di legge

che, nonostante le denunce e le condanne, vengono reiterate nei confronti delle donne spesso da parte di familiari o di persone che hanno vissuto accanto a loro. Invito, pertanto, le colleghe a far convergere lì tutti i nostri sforzi nella

di precise indicazioni che provenivano dal Governatore della Banca d'Italia, nonché dal Fondo monetario internazionale. Il Governatore della Banca d'Italia,

i risultati positivi ottenuti dagli ordinamenti che puniscono anche il cosiddetto autoriciclaggio. Tali considerazioni erano state

finalmente si accoglierebbero i rilievi formulati dal Fondo monetario internazionale del 2005, suggerendo un intervento legislativo in tal senso, anche alla luce dei risultati positivi raggiunti dagli ordinamenti di altri Paesi,

di punizione delll'autoriciclaggio. Non capisco ora questa marcia indietro rispetto ad un qualcosa che si faceva nell'interesse condiviso da parte di tutti; non capisco la necessità di collocare questa norma in un ampio testo diverso. Quale è questo testo? Stiamo parlando di riciclaggio e autoriciclaggio, di una norma che ci era stata suggerita dal Fondo monetario internazionale, dal Governatore della Banca d'Italia, dal procuratore nazionale antimafia, proposta da noi dell'opposizione, proposta dalla Commissione antimafia all'unanimità nella scorsa legislatura, fatta propria dai relatori e presentata dai relatori stessi. Ora si dice di no. Perché? Perché dobbiamo rinunciare a questo strumento di contrasto all'autoriciclaggio, che è un fenomeno particolarmente grave e impeditivo di accertamenti? Si dice che ce ne occuperemo in un altro momento. Ebbene, dato che non esistono ragioni

sono anche le mie considerazioni. Il reato di autoriciclaggio è estremamente importante e viene richiesto ai più diversi livelli, da quelli altissimi, menzionati dal senatore Li Gotti, a quelli delle forze dell'ordine in generale, per risolvere problemi che vedono non punita un'attività di riciclaggio da parte dell'autore del reato. Ciò fa sì che si creino delle zone d'ombra che non permettono di perseguire i colpevoli sotto diversi profili, non solo penali ma anche di conseguenze penali del reato, quali sequestri o confische. Conosco l'obiezione di parte della dottrina che è stata pubblicata anche recentemente su «Il Sole 24 ORE». In sostanza, questa dottrina dice con la norma sull'autoriciclaggio, per come è stata scritta dalle Commissioni riunite, si va a fare eccezione al principio consolidato del diritto penale secondo il quale il *post factum* non è punibile. punibile. L'autore del reato, quindi, è punibile solo del reato presupposto e non di questo autoriciclaggio che verrebbe da tale dottrina considerato *post factum*.

debbano, quindi, essere introdotti proprio per la fondamentale utilità della quale ho brevemente

della normativa che riguarda l'autoriciclaggio. Noi siamo fortemente e convintamente favorevoli a una riformulazione delle norme di cui agli articoli 648-*bi*s Il problema è squisitamente di natura tecnica; non esistono soltanto gli articoli de «Il Sole 24 Ore»,

quindi, come abbiamo già segnalato all'interno delle Commissioni riunite, un approfondimento tecnico specifico. Abbiamo riproposto in questa sede una soppressione dei commi 4 e 5, ma proprio per dare la la nostra convinta idea che sosteniamo la necessità di affrontare il tema del *post factum*, come giustamente diceva il senatore Boscetto, voteremo a favore

Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio le disposizioni dell'articolo 1, commi 4 e 5, del disegno di legge n. 733, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, costituiranno un autonomo disegno di legge (733-*bis*) dal titolo «Modifiche degli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale». Tale disegno di legge sarà assegnato alle competenti Commissioni parlamentari. Signor Presidente, richiamo l'attenzione del Governo e dei relatori su qualcosa che non riesco a capire.

il nostro voto contrario, la maggioranza aveva modificato gli articoli 235 e 312 del codice penale, prevedendo la reclusione da sei mesi a quattro anni nel caso in cui

per quale motivo venga tenuta ferma questa previsione con riferimento all'articolo 235 e, invece, sia stata

come era stato modificato con la previsione di sanzioni da sei mesi a quattro anni per il trasgressore all'ordine di espulsione, si riferiva

di cospirazione politica, di banda armata, di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, cioè una serie di reati gravi: per quale motivo per questo tipo di reato la maggioranza ritiene improvvisamente che debba essere abrogato il comma 2 dell'articolo 312, che era stato inserito nel luglio 2008? Di fronte a questa schizofrenica scelta, per noi incomprensibile, di fronte alla chiusura sulla modifica che si riteneva opportuna ed è condivisa, ossia irrigidire lo strumento di concessione del beneficio di sospensione della pena,

per il ripristino del reato di oltraggio, che tutela l'azione delle forze dell'ordine e l'attività della polizia giudiziaria. Già gli interventi del senatore Benedetti Valentini e del senatore Saltamartini hanno sottolineato questo fatto, che ha una valenza giuridica per le sanzioni che sono connesse all'oltraggio nei confronti degli operatori della sicurezza, ma anche una valenza di ordine morale. Dedichiamo pertanto a tutti coloro che operano

perché le leggi hanno una storia: era già arrivato quasi al voto finale nella precedente legislatura: lo abbiamo ripresentato per primi; abbiamo chiesto a questa Camera

non c'è chi non veda - e l'ultimo emendamento presentato dal Governo va in tal senso - che ci vuole una revisione della Fini-Bossi. Ci vuole una revisione della Fini-Bossi perché tutto il marchingegno non funziona.

salvare l'onore delle forze dell'ordine senza dare una lira piuttosto difendere invece la salute e la vita delle donne. Detto questo, chiediamo il voto

condividendo nel merito tutti gli emendamenti presentati che sono parte integrante del disegno di legge sullo *stalking* in esame alla Camera, confermo e ribadisco la nostra volontà di ritrovarci su posizioni condivise quando quel disegno di legge arriverà - molto presto - in Senato.

legislativo, e quindi tutto nostro. Dipende solo dalla nostra volontà politica poter votare molto rapidamente in Aula il testo che la Camera ci invierà, sul quale sono certa che maggioranza e opposizione si ritroveranno. Nel frattempo, è evidente - e questo lo dico ovviamente solo a titolo personale - che su questo emendamento che si riferisce allo *stalking* è molto forte il nostro convincimento di sostenere gli sforzi che anche il Governo sta compiendo, e cioè il ministro Carfagna.

che, nel momento in cui un ramo del Parlamento sta affrontando una questione, l'altro ramo si sovrapponga con un emendamento che passa senza l'approfondimento

Quindi, si deve dare risposta al quesito: la Camera sta affrontando o no l'argomento? Se lo sta affrontando bisogna lasciarle la possibilità di approfondirlo e di portarlo a compimento. Per tale ragione ribadisco l'invito al ritiro

ritengo che a questo punto, di fronte alle dichiarazioni di disponibilità della maggioranza e del Governo, sarebbe opportuno che quest'ultimo segnalasse all'altro ramo del Parlamento questo disegno di legge come priorità da affrontare, visto che c'è un amplissimo consenso.

fa riferimento all'articolo 444 del codice di procedura penale che concerne,in particolare, il patteggiamento della pena. Ora, siamo tutti a conoscenza del fatto che spesso, specialmente per i reati di minore gravità, si accede al patteggiamento della pena, di intesa tra pubblico ministero e persona offesa, il giudice emette la sentenza. Con l'emendamento in esame si chiede che il giudice possa subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno. crede che sia un principio fondamentale di giustizia e di equità, anche sociale, pensare anche alla tutela delle vittime del reato.

che è sicuramente inferiore al limite della sospensione condizionale. Peraltro, la vittima del reato oltre al danno spesso rischia anche la beffa perché non ottiene concretamente il risarcimento del danno subito. Per questi casi, se il Parlamento volesse veramente assicurare una tutela completa in favore della vittima, bisognerebbe subordinare la sospensione condizionale in particolare al risarcimento del danno.

Quando vengono irrogate sanzioni penali di condanna, che nella maggior parte dei casi sono di molto inferiori al limite della sospensione condizionale della pena, prima di arrivare ad un risarcimento del danno reale per i lavoratori e le vittime,

che si debba introdurre il principio del risarcimento del danno o la eliminazione delle sue conseguenze come condizione per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

dell'aspetto sanzionatorio della norma, pur importante e insostituibile, si ponga l'esigenza della riparazione o del ristoro del danno, del suo risarcimento. È quello che oggi, specialmente di fronte alle pastoie, alle lungaggini, alla causidicità della nostra giustizia, il cittadino chiede. Prima sono stati fatti alcuni esempi di fattispecie di reato, ma ne potremmo fare molti altri. Quindi, questo principio riparatorio o restitutorio, immediato e comunque posto come condizione per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è un principio al quale aderisco assolutamente sia in via dottrinaria sia in via pratica. Il problema qual è? Che si va ad introdurre un principio generale nel nostro ordinamento e poiché il Governo ci annuncia - ed è vivo il dibattito politico al riguardo - un pacchetto giustizia complessivo che andrebbe ad incidere sul processo penale e, addirittura, sul diritto penale sostanziale, riconosco che in effetti questo principio si va ad iscrivere nelle norme di sistema (userei proprio la esse maiuscola per questa parola). Quindi con assoluto spirito di attesa e di impazienza quasi, nell'aderire al principio che anche il collega Casson ha illustrato, mi sembrerebbe corretto, dal punto di vista dell'intervento legislativo, attendere attendere questa riforma complessiva di procedura, ma più ancora di diritto penale nel merito per introdurre questo principio generale. Con questo cosa voglio dire?

al nostro Governo - di cui mi permetto di richiamare l'onorevole attenzione - perché non manchi di introdurre nella riforma del diritto penale, il cui pacchetto ci viene annunciato come imminente, questo principio giuridico, e cioè che per ogni beneficio di legge - sono ormai molti, oltre alla sospensione condizionale della pena, previsti per il reo riconosciuto tale - sia inserito in via generale il sacrosanto principio della condizione dell'avvenuta restituzione o ristoro del danno o della eliminazione dei suoi effetti nei confronti della parte offesa. Quindi, aderisco alla metodologia della richiesta di ritiro in questa sede, aderendo invece nel merito alla bontà del principio, ma lo trasformo e lo enfatizzo come un preciso invito - perlomeno a titolo personale, non so se di tutta l'Assemblea, non mi prendo la libertà di dirlo - all'Esecutivo affinché nel pacchetto giustizia la riforma del penale sostanziale preveda questo questo sacrosanto principio atteso da ogni cittadino perbene.

firmataria la senatrice Della Monica e che ha come oggetto la tutela della vittima di delitti a sfondo sessuale, così come per l'altro emendamento, chiedo ai presentatori di ritirarlo perché alla Camera è già incardinato un disegno di legge sul medesimo tema. Per quanto riguarda

il Governo, per bocca del Ministro della giustizia, ha annunciato che nel Consiglio dei ministri del 23 gennaio prossimo verrà approvato il testo concernente la riforma del processo penale.

Commissione giustizia, abbiamo incardinato dei disegni di legge sul medesimo tema, nel senso della riforma del processo penale, in cui rientra chiaramente la modifica dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ma soprattutto in attesa della già annunciata presentazione da parte del Governo, e in questo caso del Ministro della giustizia, di un organico disegno di legge di riforma del processo penale.

aderire alla proposizione del suddetto emendamento perché ne condivido il contenuto, al li là del fatto che in Commissione giustizia sia pronto un disegno di legge che modifica l'assetto del codice è un'applicazione di pena e non è un'assunzione di responsabilità. Ne condivido il contenuto anche per il fatto che non è possibile che la parte lesa debba poi aderire e fare una causa civile per avere riconosciuto il danno. Questo è il motivo per il quale, al di là

lo stesso tipo di menomazione. È quindi soltanto un problema di ordine formale: non c'è niente di più, né niente di meno.

intervengo brevemente per ricordare all'Assemblea che l'emendamento 4.104 ha una storia relativamente remota. Esso infatti è parte dell'originario disegno di legge unificato elaborato nella precedente legislatura, in cui erano previste le restrizioni, contenute in questo disegno di legge, all'acquisizione della cittadinanza attraverso il matrimonio, ciò allo scopo di contrastare il fenomeno delle unioni di comodo. Tuttavia, per un'adeguata armonia e bilanciamento legislativo, erano altresì previste norme, e segnatamente quella oggetto del presente emendamento, che introducevano, seppur in maniera assai mite e temperata, una prima forma di *ius soli* nella disciplina dell'acquisizione della cittadinanza italiana. È bene sottolineare che quel disegno di legge, come questo emendamento, sono il frutto di una riflessione congiunta di cui parte importante, se non fondamentale, è l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia

il punto di vista delle amministrazioni locali, di chi cioè ha la percezione più concreta di come le istanze, soprattutto nel tema delicatissimo del rapporto tra integrazione e repressione dei comportamenti devianti, si atteggino sul territorio. La storia dell'emendamento 4.104 è questa;

con l'emendamento 4.101 intendiamo ristabilire un principio di diritto fondamentale nei rapporti con la pubblica amministrazione, vale a dire la certezza dei tempi di ottenimento del decreto di cui all'articolo 7 della legge n. 91 del 1992 e delle conseguenze che ne derivino. La proposta del Governo infatti stabilisce che per l'esito positivo dell'istanza di concessione di cittadinanza non sia intervenuta separazione personale o divorzio, scioglimento o annullamento del matrimonio alla data di emissione del decreto stesso. Come visto, i casi di ritardo dell'amministrazione sono a volte eclatanti e non vi sono, si sa, rimedi giudiziali adeguati per spingere il Ministero a pronunciarsi nei termini di legge. silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione in materia di cittadinanza, un provvedimento discrezionale della pubblica amministrazione, non rappresenta nei fatti che un ennesimo e costoso tassello per il cittadino straniero. Dunque, ancorare la situazione di fatto utile per la concessione della cittadinanza al momento dell'emissione del decreto significa esporre l'istante alla mercé dei tempi e delle inefficienze del Ministero e, comunque, rendere del tutto incerti, contrariamente a qualunque principio del diritto, il se e il quando dell'istanza a tempi futuri.

sugli immigrati, di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni e sulla quale si è manifestata una rilevante incertezza all'interno della maggioranza e del Governo. Ritengo che su una materia così seria e delicata occorrerebbe procedere senza improvvisazioni, ma poiché sulla stessa tematica il Governo è intervenuto con un nuovo emendamento all'articolo 39 che riguarda sostanzialmente questa fattispecie, chiedo al relatore di esprimere il suo parere su un accantonamento dell'emendamento soppressivo 4.108, in modo tale che si possa trattare della delicata questione in un unico momento, in un unico momento, quando esamineremo la materia su cui interviene l'emendamento del Governo che certamente, anche se non identica, è affine.

sulle richieste di chiarimenti interverrà il presidente Vizzini. Per quanto riguarda i pareri, gli

dalla disciolta federazione della ex Jugoslavia. Presso la Camera dei deputati è già incardinato un disegno di legge concernente la cittadinanza

Presidente, in ordine alla richiesta del senatore Bianco circa l'accantonamento dell'emendamento 4.108, il parere dei relatori è contrario giacché quest'ultimo si occupa di materia diversa da quella che verrà poi trattata dagli emendamenti del Governo all'articolo 39, trattandosi nel primo caso delle istanze di cittadinanza e nell'ipotesi dell'articolo 39

ha per oggetto la sicurezza e l'articolo 4 nell'attuale formulazione punta ad evitare gli aggiramenti delle norme sulla cittadinanza e gli abusi relativi all'applicazione delle disposizioni che incidono sulla sicurezza. La materia a regime viene in questo momento considerata e approfondita dalla Camera e quindi, in coerenza

si tratta di questioni assolutamente diverse, perché mentre il permesso di soggiorno è soggetto poi, qualora dovesse essere confermata l'ipotesi passata già in Commissione, ad un periodico

in base alla legislazione vigente, come noto, cade almeno dieci anni dopo l'ottenimento del primo permesso di soggiorno, in una situazione del tutto diversa rispetto a quella dell'immigrato regolare che per la prima volta riceve il titolo giustificativo della sua presenza.

Presidente, noi manteniamo l'emendamento 4.108 e ci dispiace che il del Governo ed il relatore non abbiano accettato la nostra richiesta di accantonarlo. È ovvio che si tratta di materia diversa: una cosa è la cittadinanza e altra cosa è il permesso di lavoro. Tuttavia, è ovvio anche che sono questioni strettamente connesse e nessuno può negare che siamo nell'ambito della stessa impostazione culturale, cioè si ritiene che il cittadino che acquisisce la cittadinanza italiana sulla base di un soggiorno nel nostro Paese, protratto per dieci anni o per il tempo richiesto dalla legge, a differenza di chi diventa cittadino italiano per altre ragioni debba pagare allo Stato una sorta di tassa. Non si tratta di una cifra particolarmente consistente ed è certamente *una tantum*, tantum*, ma è comunque, dal punto di vista culturale, cosa che non rientra nella nostra concezione: a qualunque titolo un cittadino entri e divenga cittadino italiano deve avere parità di trattamento. Ecco la ragione per la quale chiediamo la soppressione

gli emendamenti che abbiamo proposto ce n'è anche uno che vuole introdurre il reato di tortura in Italia, dopo anni che si porta avanti un dibattito in proposito. Non ritiriamo questo emendamento, perché i tempi legali del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241 del 1990, di concessione di cittadinanza, previsti all'articolo 3 del decreto del ossia il regolamento che attua le procedure della legge n. 91 del 1992, sono di due anni, cioè di 730 giorni. Non solo, ma dal sito ma dal sito dell'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC), che haaperto una sezione particolare relativamente all'immigrazione, abbiamo raccolto tutta una serie di testimonianze secondo le quali le procedure di fatto durano molto più tempo rispetto ai due anni previsti, arrivando a quattro o più o più anni, senza che sia stata fornita alcuna giustificazione relativamente al ritardo. Riteniamo quindi che due anni, senza che venga fornita una dettagliata istruttoria di ciò che va portando avanti l'amministrazione pubblica, costituiscano un tempo troppo lungo per questo tipo di procedure. Per tale ragione, con il nostro

visto che si tratta di una fattispecie molto specifica e piuttosto combattuta. Ci sono sicuramente situazioni di profughi degne di essere considerate perché riguardano in particolare i minorenni.

a restringere il limite della portata del nostro emendamento. Peraltro, condividiamo la valutazione della necessità di rivedere completamente l'assetto concernente anche i cittadini provenienti dalla disciolta Federazione della ex Jugoslavia.

il matrimonio dello straniero nella nostra Repubblica è già ben disciplinato in maniera organica e completa dell'articolo 116 del codice civile, sia per quanto riguarda il nulla osta che è richiesto all'autorità dello Stato straniero, sia per quanto riguarda gli atti di controllo e di verifica che sono in capo alle autorità che presiedono agli uffici dello stato civile nel nostro Paese.

gli innumerevoli sbarchi clandestini che abbiamo registrato in questo periodo, ci fanno dire che tra la quantità di parole e l'effettiva produzione di fatti vi sia un rapporto inversamente proporzionale. Per questi motivi chiediamo la soppressione dell'articolo 5.

Presidente, chiedo l'accantonamento dell'articolo 7 perché abbiamo delle questioni da risolvere sugli emendamenti e sul testo approvato dalla Commissione.

di quest'Assemblea e abbiamo lavorato anche in Commissione - su quali sono le "questioni" per le quali si chiede l'accantonamento

comportano un intervento sul piano ordinamentale per poter corrispondere le retribuzioni mensili al personale delle forze di polizia. di polizia. Data l'importanza di questo provvedimento, che potrebbe comportare un ritardo nei meccanismi di pagamento degli emolumenti, chiedo che il Governo sostenga

ascoltarmi - ci sarà ancora qualche ora per la trattazione dell'intero provvedimento e confido nella possibilità di un esame ancora più analitico del sostegno finanziario che finora non è stato ritenuto congruo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione

Presidente, poiché le richieste di accantonamento non sono questioni personali, immagino che se il senatore Vizzini richiede un accantonamento per una discussione politica, l'Assemblea, e in particolare i colleghi della Commissione che hanno lavorato con lui in modo molto serio, abbiano il diritto di essere informati sulle ragioni politiche per affrontarle e possibilmente dare un contributo per risolverle.

e gli esercenti che sono in possesso, invece, di una concessione ma non ottemperano alle prescrizioni, travalicando i confini degli spazi assegnati. La differenza ha una sua *ratio* anche nella previsione dell'articolo 20 del codice della strada: infatti, per entrambi i casi, vi è una sanzione amministrativa che permette una gradazione, consentendo la possibilità di modificare la sanzione a seconda della gravità dell'infrazione. Il secondo emendamento, invece, è volto ad evitare che vi sia confusione in materia di sanzioni che hanno a che fare con l'occupazione abusiva di suolo pubblico, perché molti regolamenti comunali già prevedono il ripristino dello stato dei luoghi. Quindi si dice che le disposizioni

l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti dei parcheggiatori abusivi, ritenendo che il comportamento di questa persone incide oltremodo in maniera negativa nei confronti della qualità della vita delle persone, rientrando nella cosiddetta È una proposta nata all'interno del tavolo sulla sicurezza creato in Piemonte, nella fattispecie a Torino. Questo emendamento intende offrire uno strumento di più pregnante efficacia nell'azione di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, la cui attività è spesso caratterizzata da comportamenti sia aggressivi sia intimidatori,

poiché gli attuali strumenti di contrasto sono di natura eminentemente contravvenzionale, sono di fatto totalmente inapplicabili e si mostrano totalmente inefficaci a debellare questo fenomeno, si ritiene opportuno che ci sia la possibilità di estendere invece a tale attività la definizione di comportamento pericoloso per la sicurezza pubblica e, di conseguenza, l'applicazione delle misure preventive previste nella vigente legislazione.

della fattispecie dell'impiego di minori nell'accattonaggio, che, da semplice contravvenzione, diviene vero e proprio delitto. Secondo noi le misure necessarie per affrontare tale fenomeno (che naturalmente esiste, nessuno vuole negarne l'evidenza) debbono essere di tipo completamente diverso e mirare molto di più all'estensione dei diritti di cittadinanza alle suddette comunità presenti in Italia ed eventualmente a politiche di integrazione sociale e culturale, nonché economica.

la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale. Abbiamo dinanzi un quadro di sfruttamento che riguarda comportamenti di genitori irresponsabili e, sotto certi aspetti, diretti a non tutelare la persona del figlio, che è posta sotto il loro diretto controllo. Vi è un aspetto però di questo delicato problema e di questa delicata pena accessoria che attiene non alla persona del genitore ma soprattutto agli effetti che si riverberano sul minore: la complessità delle situazioni familiari, che vedo sfociare anche in questo comportamento sanzionato, è tale da imporre una valutazione complessiva molto attenta.

un ascolto, cioè una decisione del tribunale dei minorenni, al fine di non perdere il contatto e la relazione con i genitori, che, sebbene rei di fatti illeciti, potrebbe essere necessaria, se non indispensabile, per lo sviluppo della vita e soprattutto dell'equilibrio del minore. Questa è la ragione fondamentale dell'esistenza nel nostro ordinamento di tutto il sistema civile e penale affidato alla giurisdizione in in favore dei minorenni. Pertanto, prima di irrogare una sanzione che vada ad incidere non tanto e non solo sulla persona del reo ma soprattutto sulla persona del minore, pensiamo sia indispensabile nell'interesse superiore del minore che il tribunale

alla censura e alla repressione di questa forma di illecito, cose che noi condividiamo, ma che mira esclusivamente a salvaguardare l'equilibrio e l'interesse superiore del minore. colleghe e colleghi, gli emendamenti 12.0.100 e 12.0.300 tendono ad introdurre l'assistenza pediatrica per i bambini immigrati i cui genitori non siano in regola con il permesso di soggiorno. Sono emendamenti che modificano l'assistenza sanitaria nel senso di dare stabilità e continuità al diritto alla salute dei bambini.

siano previste una serie di cure essenziali. Tra queste cure essenziali, al capoverso *b)* si parla anche della tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo. Anche se la 5a Commissione non ha segnalato problemi di copertura - perché non ce ne sono in quanto la voce di bilancio è una voce di carattere generale

Quella potrebbe essere, invece, la sede più opportuna per dare una risposta adeguata ai problemi che vengono sollevati e per vedere se dipendono da una legislazione nazionale o da linee di indirizzo

sanzione e all'inasprimento della sanzione per chi utilizza i minori nell'accattonaggio, ma con questo emendamento chiediamo di introdurre un'ipotesi aggravata per chi utilizzi minori di tre anni (una delle ipotesi più ricorrenti nello sfruttamento dei minori in questo campo).

minori stranieri segregati in questi centri. E poiché il nostro ordinamento, in ossequio alle Convenzioni internazionali, prevede che i minori stranieri irregolari non solo siano inespellibili, ma devono essere trattati dal nostro ordinamento alla stregua dei minori italiani che si trovano in condizioni di disagio e quindi avviati presso centri e strutture adeguati che siano nelle condizioni di poterli assistere, è evidente che, ad esempio, il caso dei 150 giovani minorenni minorenni segregati a Lampedusa (parte dei quali sembrerebbe siano stati già trasferiti) è un caso che non fa onore al nostro Paese. Credo che gli interventi che vanno nel senso di rafforzare la tutela dei minori irregolari che arrivano nel nostro Paese e che si trovano, soprattutto se non accompagnati, in condizioni di assoluto disagio e solitudine debbano essere accolti. Ritengo che non possa neanche far velo l'eventuale reperimento di una copertura diversa,

che cerchiamo di garantire ai minori italiani, forse facciamo un lavoro migliore ed evitiamo alcune passerelle indecenti come quella di Lampedusa.

chiedo a dodici colleghi il sostegno per la verifica del numero legale.